Signor Presidente, senatrici e senatori, la situazione in Venezuela merita tutta la nostra attenzione e preoccupazione.

di italiani e anche cittadini italiani presenti in Venezuela. Siamo sempre stati fautori di una risposta europea a questa crisi, come peraltro alle altre crisi con le quali ci confrontiamo nello scenario mondiale. Riteniamo che sia giusto perseguire - è quanto l'Italia ha sempre fatto e quanto sta facendo il Governo - una soluzione pacifica e democratica per questo Paese a noi così vicino. Se mi consentite, passo a una ricostruzione degli eventi che hanno portato alla situazione Nel maggio dello scorso anno si sono svolte elezioni presidenziali anticipate, che hanno portato alla riconferma riconferma dell'attuale presidente, Nicolás Maduro. Queste elezioni sono state giudicate dalla comunità internazionale e dagli osservatori come non libere e non trasparenti. Di conseguenza, la legittimità dell'attuale Presidente del Venezuela ne è uscita fortemente inficiata. I fattori che hanno determinato questo giudizio possono schematicamente riepilogarsi nei seguenti: la partecipazione degli elettori al voto è stata bassa - inusualmente bassa - in un Paese dove normalmente è elevata; ci sono state delle decisioni giudiziarie quantomeno discutibili, che hanno portato a escludere svariati esponenti dell'opposizione dalla competizione elettorale; vi sono state numerose denunce di irregolarità il risultato non è stato riconosciuto dalla coalizione di opposizione, né dall'Organizzazione degli Stati americani,

di nuove elezioni, purché libere e trasparenti. Nel giugno dello scorso anno, di fronte a un'assenza di progressi, a livello di Unione europea è stato approvato un pacchetto di misure sanzionatorie cosiddette individuali, perché colpiscono singole persone: 11 esponenti dell'attuale regime di Governo in Venezuela sono stati ritenuti responsabili e, quindi, sanzionati per violazioni che che riguardano i diritti umani e le regole democratiche. L'obiettivo delle violazioni era mantenere una forma di stimolo, di pressione, affinché si procedesse a un dialogo tra le forze politiche venezuelane e possibilmente a un ristabilimento pieno del quadro di legittimità democratica. In realtà, è accaduto che, il 5 agosto sempre del 2018, c'è stato un presunto attentato in presenza del presidente Maduro e questo ha causato una serie di interventi che sono stati portati avanti nei confronti delle opposizioni, che venivano indicate dal regime come colpevoli. Ciò, naturalmente, ha comportato a sua volta un'ulteriore reazione a livello di comunità

- hanno preso una decisione molto rara nelle relazioni internazionali, vale a dire il deferimento del Venezuela alla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità. un atto d'accusa di una gravità all'evidenza molto forte. L'Unione europea, dal canto suo, con il pieno sostegno e la partecipazione dell'Italia, ha sempre insistito su cinque punti che - sempre nel tentativo di essere chiaro - mi permetto di schematizzare: il primo, il pieno ripristino e il rispetto dei poteri dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta in elezioni giudicate valide dalla comunità internazionale e dagli osservatori; il secondo, l'indizione di nuove elezioni presidenziali credibili (il punto costante di questa vicenda nella posizione dell'Unione europea); il terzo, il rilascio di tutti i prigionieri qualificabili come prigionieri politici; il quarto, la piena garanzia della libertà di espressione e di informazione (quindi, siamo alle libertà basilari); il quinto, l'apertura di appositi corridoi umanitari per consentire l'afflusso di aiuti internazionali a favore della popolazione. Vi ricordo che uno dei tre elementi gravi di questa situazione è proprio l'emergenza sociale che tocca strati diversi della popolazione venezuelana. Questo è peraltro l'ulteriore sviluppo degli ultimi mesi: una vera e propria crisi di rifugiati, persone che lasciano il Venezuela per cercare rifugio e situazioni migliori in Paesi confinanti. è intervenuta a questo riguardo - lo segnalo come esempio particolare - con un finanziamento di 500.000 euro all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e si è fatta promotrice - a fine ottobre 2018 - di un inizio di fase esplorativa dell'Unione europea, insieme a Paesi latino-americani, per cercare di facilitare il dialogo tra Governo e opposizione. Arriviamo agli sviluppi più recenti. Il 10 gennaio il presidente Maduro si è insediato - nella situazione di non piena legittimità democratica di cui abbiamo già detto - per il suo secondo mandato. Gli ambasciatori degli Stati dell'Unione europea non sono stati presenti alla cerimonia cosiddetta di insediamento, per decisione evidentemente coordinata a livello di Unione. Successivamente sono state assunte delle iniziative, da parte del Governo, per restringere la

fuori da questo supporto Messico e Uruguay, che hanno espresso una posizione comune per un negoziato fra Governo e opposizione in Venezuela. sul fronte opposto di sostegno al presidente Maduro troviamo Cuba, Russia, Cina, Turchia, Nicaragua e Bolivia. Ci sono state espressioni di preoccupazione da parte della Santa Sede e, per quanto riguarda l'Unione europea, al Consiglio affari esteri del 21 gennaio è stato discusso, ancora una volta, lo stato della situazione in Venezuela. Un piccolo gruppo di Paesi (Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi) ha fatto una dichiarazione insieme - sempre il 21 gennaio - per rendere più veloce la costituzione del cosiddetto gruppo di contatto internazionale, che dovrebbe riunire Paesi dell'America latina e Paesi europei, per cercare di ristabilire i fili del dialogo - o del negoziato, se vogliamo chiamarlo così - tra Governo e opposizione e, possibilmente - quanto negli intenti dei Paesi europei e dell'America latina - portare a un ristabilimento pieno della legittimità democratica. Successivamente, il 23 gennaio scorso c'è stata una prima dichiarazione a 28 - tutti gli Stati attualmente membri dell'Unione europea - contro l'uso della forza da parte della polizia e a sostegno della libertà di manifestazione, perché era in atto una repressione delle manifestazioni contrarie al Governo. Arriviamo infine agli ultimissimi avvenimenti. Tra venerdì 25 e sabato 26 gennaio è stata discussa, a livello di contatti intensi tra gli Stati membri dell'Unione europea, una dichiarazione comune - alla

repressione e il sostegno all'Assemblea nazionale, organo democraticamente legittimato. Come terzo elemento, vi è un pressante appello per la convocazione di elezioni, con un annuncio da farsi già nei prossimi giorni, rispetto a questo sabato 26. Come quarto elemento, nel caso in cui non ci dovesse essere detto annuncio e non si dovesse procedere verso nuove elezioni, i Paesi dell'Unione europea si riservano ulteriori iniziative. Viene menzionato come esempio, con la terminologia «ivi inclusa», la questione del riconoscimento di una diversa *leadership* nel Paese, secondo quanto previsto dall'articolo 233

parte - ripeto - Paesi latino-americani e Stati membri dell'Unione europea. Alcuni degli Stati membri dell'Unione europea - 6 su 28 specifico, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Portogallo - hanno ritenuto di dover esprimere una posizione più netta rispetto alla posizione comune di cui vi ho detto. In particolare, hanno indicato

appoggio al Presidente dell'Assemblea e alla sua attuale posizione di autoproclamazione, ai sensi della Costituzione venezuelana, come capo del Governo. riguarda la posizione italiana, ci riconosciamo pienamente nella dichiarazione dell'Unione europea, in particolare l'ultima, quella di sabato 26 gennaio; una posizione che ribadisce un obiettivo di risultato: arrivare a arrivare a elezioni libere, democraticamente riconoscibili e trasparenti per il Presidente della Repubblica. Ci riconosciamo anche nella indicazione di un termine di giorni entro i quali debba arrivare l'annuncio delle nuove elezioni, anche se nella dichiarazione europea questo termine non è cifrato, a differenza di ciò che, invece, avviene nella dichiarazione dei sei Paesi di cui vi ho detto. Teniamo presente che la situazione in Venezuela si può definire, con un termine neutrale, fluida; è una situazione tesa, in cui non dobbiamo dimenticare che la priorità deve essere quella di evitare

L'obiettivo fondamentale della linea del Governo è restituire la scelta democratica al popolo venezuelano. Su questo non ci devono essere dubbi. di arrivare a nuove elezioni, libere e trasparenti, pienamente riconoscibili dalla comunità internazionale, non è assolutamente da mettere in dubbio. Pensiamo che occorra lavorare per favorire siffatto processo nel migliore dei modi. Rispetto a questo, rimaniamo impegnati e troviamo che la costituzione del gruppo internazionale di contatto rappresenterebbe un passo importante, perché permetterebbe di avere un gruppo permanente, permanente, nella misura in cui sarebbe stabile rispetto all'attuale crisi, che può fungere da stimolo e da osservatore, anche per rendere note pubblicamente eventuali derive.

Siamo fortemente impegnati per gli italiani e i cittadini venezuelani di origine italiana che si trovano nel Paese, così come riserviamo particolare attenzione alle nostre aziende. Abbiamo preso alcune misure puntuali, che cito brevemente a titolo di esempio e naturalmente siamo a disposizione per dare maggiori dettagli. Abbiamo provveduto a intervenire sull'integrazione del minimo pensionistico. Tenete conto che vi è un'emergenza sociale: possono sembrare misure

per chi si trova in Venezuela e con un piano straordinario di assistenza ai gruppi più vulnerabili, stanziando per i nostri compatrioti più bisognosi che si trovano in Venezuela la somma di circa due milioni di euro. Abbiamo provveduto a stabilire un fondo in grado di provvedere alla fornitura diretta di medicinali che non sono più reperibili sul mercato locale e, sempre nell'ordine di questi esempi, abbiamo sospeso l'adeguamento automatico della tariffa percepita per i servizi consolari, che viene adeguata automaticamente alla svalutazione della moneta venezuelana. Questa è una misura importante, perché la svalutazione ha raggiunto dei ritmi di grande rilievo. I nostri servizi consolari e di ambasciata operano a pieno ritmo, in assistenza agli italiani e ai cittadini di origine italiana. Abbiamo rafforzato le misure

ha l'obiettivo di fornire il massimo delle informazioni, vengono fornite tutte le informazioni necessarie. Un'ultima parola pronuncio sul caso della cittadina italo-venezuelana Laura Beatriz Gallo, Gallo, attivista dell'opposizione, che è stata tratta in arresto nel corso delle manifestazioni di protesta del 23 gennaio scorso. La nostra ambasciata ha preso tutte le informazioni e sta fornendo assistenza, in particolare per verificare le sue condizioni di salute e di detenzione. Siamo in contatto con i familiari e con i legali, naturalmente, come sempre accade quando ci sono queste situazioni di difficoltà per gli italiani all'estero. La situazione processuale è la seguente: il giudice aveva disposto una una libertà condizionata, c'è stata un'opposizione in appello da parte della pubblica accusa e ora si deve pronunciare il giudice di appello. Questo è il quadro, mi auguro utile. Avremo ulteriori aggiornamenti sulle posizioni europee a valle della riunione di cui vi

agli italiani in Venezuela, che sono sicuramente in questo momento - come ci hanno segnalato già da qualche giorno in contatto con questa Aula in modo materiale, nel senso che stanno seguendo il dibattito che avviene qui al Senato. Lo hanno aspettato con ansia. Il Governo finalmente si è presentato, dopo quattro o cinque giorni dalle nostre richieste, secondo me tardivamente. Vorrei anche dire a quegli italiani che tanti di coloro che sono presenti in quest'Aula saranno sabato in piazza con la comunità venezuelana in Italia, a manifestare per la libertà di quel Paese. Lo voglio dire e voglio sgomberare il campo da un problema: tutti voi sapete in quest'Aula, per la mia lunga militanza, che sono considerato quasi sempre un sempre un mediatore, anche in eccesso, una persona che cerca e rifugge gli estremismi. È vero, sono così, è la mia natura e non solo la mia vocazione politica. E sono anche uno che non fa mai delle polemiche personali. infatti dire al ministro Moavero Milanesi, che stimo, che mi rendo conto della sua situazione e vorrei sgomberare il campo anche dal fatto che le considerazioni che farò siano rivolte personalmente al Ministro. Siamo tutti troppo intelligenti non capire che il Ministro siede in un Governo dove, sul tema dell'Afghanistan, il Ministro della difesa ha spiegato che non era tenuto ad avvertire il Ministro degli affari esteri.

quello che il Ministro degli affari esteri ha detto adesso, che è una comunicazione burocratica ineccepibile sulla burocratica posizione che il Governo italiano ha assunto, che peraltro è stata burocraticamente anticipata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che qualche ora fa - è su tutte le agenzie - ci ha spiegato che noi siamo che noi siamo per il dialogo; che noi siamo per la pace in Venezuela, e che noi vogliamo che le parti dialoghino tra di loro. Guardate: è molto difficile non essere d'accordo con questo. *(Applausi Il problema vero è che questo dialogo si è ricercato da anni. Il Vaticano ha fatto in prima persona una mediazione chiamando al tavolo tutti, e tutti hanno capito che il dialogo serviva unicamente a Maduro per prendere tempo e reprimere brutalmente l'opposizione in quello che è diventato un regime narcotrafficante, perché i collegamenti tra il traffico della droga e il regime venezuelano

abbiano espresso una posizione univoca. Io vi dico sinceramente che non è vero che il Governo italiano non si sia espresso. No, perché, se noi diciamo che questa comunicazione burocratica non è chiara, sbagliamo: è chiarissima.

«Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di Maduro, fondato su violenza, paura e fame. Quanto prima cade, senza ulteriori scontri, meglio è». Io speravo che almeno in questa circostanza, visto che Salvini conta molto nel Governo, avesse impresso questa linea al Governo italiano, che è la linea che hanno espresso non alcuni Paesi che non hanno interessi in Venezuela. Anche in questo, per favore, non siamo così ipocriti da dire che noi non prendiamo posizione per paura dei nostri connazionali. I nostri connazionali in Venezuela oggi vogliono che prendiamo posizione. La Spagna mi risulta che non abbia meno connazionali di noi in Venezuela. E io devo ringraziare il Governo spagnolo, quello francese, quello del Regno Unito, quello dei Paesi Bassi*,* che hanno con coraggio assunto una posizione. Noi abbiamo una posizione; non è vero che noi non l'abbiamo. Noi abbiamo una posizione chiarissima: il Governo italiano è per una equidistanza tra Maduro e l'Assemblea legislativa. il Governo italiano ci spiega che devono dialogare; che i due ragazzi che litigano si mettano al tavolo, perché per noi ci sono il Presidente e il Parlamento; noi non sappiamo da che parte stare; sappiamo che devono dialogare. No, no, i conti non tornano. Io so da che parte stare, il Gruppo per le Autonomie sa da che parte stare: noi scegliamo l'unico organismo legittimato dal voto popolare, quello vero, che è l'Assemblea legislativa. *(Applausi dai solidali con i nostri colleghi venezuelani che sono stati privati dello stipendio, che sono stati privati della sede. Se non Se non vi è chiaro, vi vorrei dire che il regime ha provveduto anche a tagliare la luce, il gas e tutto il resto all'Assemblea nazionale venezuelana. Almeno per solidarietà tra parlamentari, io credo che noi dovremmo esprimerci con chiarezza su questo. E invece noi scegliamo l'equidistanza. Colleghi, dal Ministro siamo tutti d'accordo. Avete visto che anche Maduro dice che occorre fare le elezioni. Oggi Maduro ha detto di essere d'accordo con la richiesta di fare elezioni garantite democraticamente,

e spero che il Governo italiano cambi posizione. Spero che il Governo italiano decida da che parte stare. Spero che il Governo italiano scelga di stare dalla parte di coloro che oggi sono in piazza e sono affamati da un regime illiberale e dispotico. Spero che il Governo italiano esca dalla stucchevole idea dell'equidistanza come se ci fossero due parti egualmente legittimate moralmente e democraticamente. No! Non sono uguali. Non sono uguali perché da una parte c'è il bene; c'è una politica che comunque cerca di lavorare nell'interesse della gente e rischia in prima persona per affermare le proprie idee e, dall'altra parte, c'è un regime che sta in piedi con i militari. E sapete perché i militari tengono i piedi questo regime? Sono compromessi fin sopra la testa con i traffici, non ultimi i narcotraffici, ormai completamente connessi con il regime venezuelano. Questa è la realtà. Io non sono un pericoloso estremista che cerca di andare in giro. Sono una persona obiettiva che in gran parte, obiettiva che in gran parte, con questo discorso, è in connessione con tutte le persone che conoscono la situazione del Venezuela e che hanno, in questi anni, seguito attentamente la situazione. Cari colleghi, è un'occasione mancata per l'Italia, l'ennesima.

Onorevole ministro Moavero Milanesi, la ringrazio per aver informato quest'Assemblea sui propositi del Governo rispetto alla crisi venezuelana. Abbiamo ascoltato con grande attenzione le sue parole e vogliamo credere che esse rappresentino davvero la posizione del Governo. Dico questo perché nei giorni scorsi, come spesso accade, diversi esponenti della maggioranza hanno espresso posizioni diverse, in certi casi addirittura contraddittorie. Io penso che la politica estera dell'Italia meriti un comportamento più serio, maggiore prudenza nelle dichiarazioni e una linea condivisa almeno a livello di Governo. Non parliamo poi delle quasi dichiarazioni di guerra a Germania, Francia e Olanda, ma soprattutto di quelle sull'impegno dei nostri militari che non possono e non devono essere esposti a maggiori rischi per le beghe di una maggioranza traballante. Voglio approfittare di questa occasione per far giungere al Presidente Conte la mia sincera solidarietà. Piuttosto che governare il Paese, il Presidente del Consiglio sembra costretto a passare la maggior parte del suo tempo a riconciliare le litigiose fazioni della sua maggioranza o a proporsi come scudo per responsabilità altrui. Seguiamo con apprensione l'evoluzione di una situazione di grande tensione: l'aggravarsi del braccio di ferro tra Nicolás Maduro e Juan Guaidó sta portando il Paese nel caos, mentre il popolo venezuelano è già profondamente sfiancato da condizioni economiche e sociali davvero drammatiche che lei stesso ha illustrato, con carenze di cibo, di medicine e di acqua, con decine di morti a seguito delle manifestazioni di protesta. Riteniamo che a di concerto con i Paesi dell'Unione europea e in conformità con il diritto internazionale, debba promuovere una forte iniziativa diplomatica utile a evitare che su questa evitare che su questa crisi si consumi uno scontro di natura geopolitica e geoeconomica che nulla ha a che fare con la vera urgenza di queste ore: evitare innanzi tutto una guerra civile e scongiurare spargimenti di sangue, nel supremo interesse di tutti i cittadini venezuelani, molti dei quali di origine italiana.

Noi di Liberi e Uguali crediamo che la comunità internazionale debba accompagnare questa fase attraverso osservatori internazionali che vigilino sul corretto svolgimento di nuove elezioni da convocare il prima possibile, attraverso il negoziato e la diplomazia con tutti i mezzi possibili, evitando che gli *ultimatum* si risolvano in occasioni di violenza fratricida. Come opposizione, sosterremo lealmente il Governo italiano in questa prospettiva e contestualmente chiediamo a lei, ministro Moavero Milanesi, di riferire tempestivamente al Parlamento le ulteriori iniziative che ella vorrà intraprendere

avere una tardiva, confusa e approssimativa informativa. Nel frattempo, a noi tutti sono arrivate centinaia, commoventi richieste d'aiuto da parte della nostra comunità in Venezuela. Due milioni di cittadini italiani - o oriundi italiani

Quella gente aspettava dal Governo della Patria d'origine una chiara presa di posizione. In questa settimana, invece, secondo il giornale più vicino al Governo, «il Fatto Quotidiano», l'Italia ha espresso quattro diverse posizioni. La prima posizione è quella da lei ribadita in quest'Aula,

che ha più connazionali in Venezuela di chiunque altro, è al seguito dell'Unione europea. In secondo luogo, lo stesso giornale parla di Salvini contro Maduro. Finalmente, dopo il primo giorno, in cui la Lega è rimasta imbarazzata e silente, senza prendere posizioni in quest'Aula, l'ha fatto il ministro dell'interno Salvini, e in maniera netta, contro il dittatore Maduro, a capo di una giunta e di un regime militare che si reggono anche sul narcotraffico. Quanto di peggio vi possa essere al mondo in questo momento.

Una quarta posizione - lo dice lo stesso giornale - è stata espressa dal *Premier*, essendo in mezzo a tutti gli altri. Aggiungo, signor Ministro degli affari esteri, che una quinta posizione è stata espressa pochi minuti fa

dice esattamente un'altra cosa. Nel comunicato ufficiale espresso dal Gruppo dei senatori del MoVimento 5 Stelle pochi minuti fa in un'agenzia, infatti, è stata espressa una quinta posizione poco prima che lei parlasse, che è la posizione della evidentemente avrà anch'essa milioni di connazionali in Venezuela e che, a differenza di quello che pensano le popolazioni dell'America latina (brasiliani, argentini, cileni, cileni, colombiani e tutti gli altri o quasi tutti gli altri), esprime un'altra posizione, perché la Grecia è molto vicina a quel Paese, ne sa molto di Venezuela, più della Spagna, più di noi, più degli americani, più dei venezuelani. Siamo quindi già a cinque diverse posizioni in vista del vertice di domani, in cui non si capisce cosa lei dirà a nome dell'Italia. E non si capisce il momento di estrema gravità, in cui a noi appare chiarissima la situazione: da una parte c'è un regime militare che si regge sul terrore. Secondo le Nazioni Unite, già in questa settimana di silenzio e latitanza da Ponzio Pilato del Governo italiano, ci sono stati 40 morti, 850 arresti (700 solo nella giornata di mercoledì scorso). Ci sono video che mostrano le torture e gli assassinii perpetrati dalla polizia segreta venezuelana;

le borgate di Caracas, che tanto avevano sperato nel regime di Chavez e che oggi sono piombate nel buio di Maduro. C'è un regime militare che è stato eletto in un'elezione

La gravità è questa. Da una parte vi è un regime intollerante, l'elezione di Maduro che è stata dichiarata una farsa; e dall'altra parte vi è un'Assemblea nazionale liberamente eletta che, in base alla Costituzione venezuelana e al diritto internazionale, elegge un Presidente *ad interim*, sia sulla base del diritto venezuelano (articolo 233 della Costituzione) sia sulla base del diritto internazionale. Non c'è dubbio da che parte stare.

né con la comunità internazionale, e nemmeno col popolo italiano, che ha molti parenti in Venezuela. *(Commenti del senatore Ferrara).* Dall'altra parte, c'è un Governo eletto da un Parlamento liberamente scelto dagli elettori. Cosa ha risposto Maduro? Lei non ce l'ha detto in quest'Aula. Maduro ha risposto già oggi alle richieste della comunità internazionale, dicendo che resterà in carica fino al 2025 - si è fatto rieleggere fino al 2025 semmai scioglierà l'Assemblea nazionale per eleggerne un'altra. La risposta c'è già stata. Ora tocca all'Europa e toccherebbe anche all'Italia - prima dell'Europa e non dopo l'Europa, non coprendosi con l'Europa, ma scoprendo il proprio volto di Paese e di Nazione - dire cosa pensa. Noi crediamo che l'Italia debba dire soltanto una cosa: quello che chiedono gli italiani in Venezuela, cioè garantire la loro libertà e la loro sopravvivenza e per la loro libertà e la loro sopravvivenza ci vogliono elezioni libere e democratiche garantite dalla comunità internazionale; elezioni presidenziali (che sono quelle illegittime),

siamo l'Italia - più forti sono i diritti degli italiani che stanno in Venezuela e più forti sono i diritti dei venezuelani che guardano all'Italia come madrepatria. Per questo crediamo che il suo intervento sia stato giustificato

con un'intensità senza precedenti e che avevano cambiato il quadro politico in Venezuela. Purtroppo non è stato possibile per le evidenti difficoltà di una maggioranza mai divisa come in politica estera: lo abbiamo visto in questo caso, così come nel caso delle missioni in Afghanistan. Serve un chiarimento io penso che non basti un'informativa; credo che servano delle comunicazioni, con delle risoluzioni sulla politica estera, perché la nostra preoccupazione è che la politica estera italiana stia cambiando radicalmente. Faccio il primo esempio concreto. La comunità italiana in Venezuela, una delle più importanti in America latina, si aspettava una risposta chiara, netta e di vicinanza dal Parlamento, che parlasse con una voce unica; questa voce non c'è stata e questo è l'elemento più grave. Parliamo di un Paese che ha conosciuto negli ultimi anni un innalzamento del 10 per cento della mortalità infantile, un'inflazione a tre cifre, una svalutazione del 95 per cento in nome del sovranismo, con una nuova moneta che ha portato ad incrementare il costo delle importazioni - lo sanno bene i nostri italiani - e dove trovare delle medicine è maledettamente complicato. Menomale

sappiamo distinguere il lavoro prezioso che fa la diplomazia per stare vicino alla nostra comunità italiana rispetto alle dichiarazioni dissennate dei *leader* della maggioranza che governa in questo momento il nostro Paese. Lo dico perché noi rischiamo di abbandonare la comunità internazionale, internazionale, la comunità delle democrazie liberali: è questo il principale rischio che vedo in questo momento, di non stare dalla parte di chi ha patito in questi anni la dittatura di Maduro. Parliamo di tre milioni i *leader* dei principali partiti di opposizione - penso a Volontà Popolare - sono stati arrestati o sono in esilio o hanno chiesto asilo nelle principali ambasciate dei Paesi latino-americani. Credo dunque che, davanti ad un episodio come quello che è accaduto nelle settimane scorse,

non voleva dire riconoscerlo; voleva dire che noi stiamo dalla parte delle democrazie liberali, stiamo con la comunità internazionale che ha deciso di condannare quegli eventi. *(Applausi dai Gruppi* *PD e* *Aut del nostro protagonismo e della solidarietà all'interno dell'Unione europea. Mai come con il Venezuela si era misurata la capacità dell'Unione europea di parlare con una voce sola. È vero o non è vero, signor Ministro, che, dopo le elezioni del maggio 2018, elezioni contestate con forza dall'Unione europea per l'assenza di osservatori internazionali, vi eravate trovati al Consiglio affari esteri Consiglio affari esteri e avevate detto in maniera netta che bisognava prendere misure restrittive, mentre al contempo la Russia - che sembra essere diventata un punto di riferimento di una parte della maggioranza - riconosceva Maduro, gli faceva i complimenti e lo invitava al Cremlino? È vero o non è vero che a dicembre, quando lei ha appoggiato con il

E nel momento in cui, a gennaio, la Mogherini riconfermava la sua preoccupazione per la situazione in Venezuela, «Reuters» e «The Guardian» pubblicavano articoli in cui dicevano che mercenari russi legati al gruppo Wagner arrivavano al fianco di Maduro in Venezuela. Davanti a questa situazione così maledettamente complicata noi dobbiamo dire da che parte stiamo; non si può tentennare: o si sta dalla parte di Russia, Cuba e dei loro amici o si sta dalla parte della comunità internazionale e delle democrazie liberali. Conosco il lavoro che viene fatto al Consiglio affari esteri e il lavoro che fa lei come Ministro, ma - non me ne voglia ne voglia - nella costruzione e nella definizione degli elementi essenziali della politica estera incidono di più le dichiarazioni dei principali *leader* della maggioranza. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza, ed è stato quello il momento di frattura fondamentale che ha aperto una nuova fase che la comunità internazionale ha colto, perlomeno i principali Paesi democratici: in testa l'Unione europea con la Francia, la Spagna e la Germania, e dovevamo esserci noi a costruire quella posizione comune. Ebbene, davanti a quel tentativo di costruire e aprire una nuova fase, l'Italia è stata silente. Anzi, no, non è stata silente: magari fosse stata silente. invece sentito voci diverse: da una parte, abbiamo sentito Salvini dire subito che era dalla parte di Trump - perché dire dalla parte dell'Unione europea evidentemente gli fa fatica; è troppo e, dall'altra parte, il nuovo capo politico del MoVimento 5 Stelle Di Battista, onnipresente in televisione, ha definito la posizione dell'Unione europea, che sarebbe stata avallata da Salvini, una «stronzata megagalattica»:

del presidente del Consiglio Conte di questa mattina: ha parlato di elezioni libere e democratiche e ha detto che non c'è bisogno di investiture. Penso che in questo momento le posizioni ambigue e gli equilibrismi non siano sinonimo di un'attenzione equilibrata o di un tentativo di mediazione, ma rischino di essere una vicinanza pericolosa a un regime repressivo, e noi abbiamo il dovere di dire con chiarezza da che parte stiamo.

anzitutto esprimo la mia preoccupazione per quanto sta accadendo in questi giorni in Venezuela. La situazione attuale è la conseguenza di un pesante conflitto istituzionale tra i poteri dello Stato venezuelano. Gli equilibri tra potere esecutivo e potere legislativo, infatti, sono compromessi a causa di una consolidazione dei rapporti tra Governo e Tribunale supremo di giustizia, che ha portato quest'ultimo - nel nel marzo 2017 - a dichiarare nulli gli atti dell'Assemblea nazionale per evidenti ragioni politiche e ad affidare le prerogative parlamentari al capo del Governo. L'autoproclamazione del capo dell'opposizione, nonché *leader* dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó, è quindi solo l'ultimo atto di uno scontro che mostra una democrazia ferita e un popolo tutt'altro che libero di esprimere la propria sovranità. La qualità di un ordinamento democratico dipende dal rispetto, da parte delle istituzioni, della libera volontà popolare e cioè dal saper accettare la sconfitta elettorale e dal rispettare l'opposizione, perché necessaria affinché sia data voce a tutti i cittadini. In questo difficile scenario vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà al popolo venezuelano e soprattutto ai nostri concittadini che vivono il nostro impegno, come Paese democratico, dovrà essere indirizzato urgentemente a sostegno del ripristino della democrazia e dei giusti equilibri istituzionali, nel rispetto della dignità e della sicurezza del popolo venezuelano.

cui è difficile approvvigionarsi di cibo e di acqua. I farmaci si comprano al mercato nero. Riceviamo dei messaggi: le colleghe Minuto, Lonardo e altri ci fanno vedere i messaggi che ricevono da persone che sono lì.

che, pochi decenni fa, era tra i più ricchi del mondo e che ha tutt'ora le potenzialità per essere tra i Paesi più ricchi, con un sottosuolo ricchissimo e una struttura economica che era forte. Oggi c'è invece un'inflazione

Dopo un anno e più di situazione insostenibile, dopo otto mesi dalle elezioni farsa del Presidente della Repubblica e dopo che sono stati tagliati la luce, l'acqua e ogni tipo di supporto all'Assemblea nazionale, il presidente Guaidó, con il consenso dell'Assemblea, ha applicato la Costituzione del Venezuela, che all'articolo 233 stabilisce chiaramente che, in mancanza del Presidente - e un Presidente eletto con elezioni farsa non è un Presidente il Presidente dell'Assemblea nazionale assume provvisoriamente il ruolo di Presidente della Repubblica per garantire di arrivare a delle elezioni. Signor Ministro, dopo sei giorni e dopo aver fatto comunicati sempre

come posizioni parimenti ammissibili, quella del presidente Maduro e quella del presidente Guaidó, se accettiamo che il Parlamento venga esautorato a beneficio di un organo nominato da un signore che è stato eletto tramite elezioni farsa, se lo accettiamo all'estero, c'è il rischio che un giorno lo si accetti anche nel nostro Paese. Noi difendiamo la libertà dell'Italia, difendiamo la libertà dei venezuelani e soprattutto difendiamo

il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha annunciato di essere in costante contatto telefonico col presidente Juan Guaidó; io avrei voluto ascoltare qualcosa del genere anche da lei o dal Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Evidentemente invece si scelgono altre vie. Domani verrà di nuovo affrontato il tema del Venezuela dal Parlamento europeo, che ha parecchie altre cose da fare, però ha trovato il tempo. Noi, in sei giorni, invece, riusciamo solo ad avere una comunicazione, senza poter esprimere un voto. il Parlamento europeo voterà delle mozioni, tra le quali penso che passeranno sicuramente quelle del Partito Popolare Europeo, che chiedono esplicitamente il riconoscimento

(SVP-PATT, UV))*. Questo ci copre di vergogna, in particolare di fronte ai nostri connazionali che soffrono in Venezuela e che hanno il coraggio di opporsi a un regime

di evidenziare che si tratta di una disponibilità costante e soprattutto seria, nel senso che gli permette di arrivare in Aula con una posizione politica certa, analitica e compiuta, checché ne dicano i nostri oppositori. Il MoVimento 5 Stelle sostiene

della riconciliazione nazionale nel Venezuela e della soluzione politica e diplomatica e soprattutto nel chiedere con forza all'Unione europea europea e all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di impegnarsi, finalmente e concretamente, in politica estera europea. Ci sembra, infatti, che finora non lo abbia mai fatto. Abbiamo appreso dalle sue parole che sulla crisi venezuelana il Governo italiano conferma di aver scelto una posizione responsabile, in linea anche con quanto espresso pochi giorni fa da Papa Francesco; credo che questo sia un punto da sottolineare. La crisi venezuelana, cari signori, non è una crisi dell'ultim'ora, come volete farci credere; è solo l'ennesima *escalation* di un contesto geopolitico caratterizzato da una condizione di instabilità interna che dura da almeno un ventennio. Nel 2015 questa crisi si è acuita enormemente, anche purtroppo grazie al calo del prezzo del petrolio; una parola che nessuno di voi però ha nominato in quest'Aula. *(Applausi dal il prezzo del barile crollò nel 2015 da 100 dollari a circa 40 dollari; questo ovviamente ha condotto il Paese in un'inesorabile crisi, anche economica.

a fronte di una grande crisi sociale, ci sia anche una grave crisi costituzionale, che vede appunto la Carta costituzionale venezuelana forzata e interpretata da tutti gli attori a proprio favore, traendone

destabilizzazioni, spargimenti di sangue e guerre, che altro non fanno se non creare altro caos e violenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chiaramente noi riteniamo che il Governo italiano debba essere legato responsabilmente alle sorti dei nostri connazionali, ma non solo, quindi anche al popolo venezuelano (ricordo che ci sono 150.000 italiani residenti e oltre 2 milioni di italo-venezuelani), nel fornire nel fornire - e questo il Ministro ce l'ha raccontato - un sostegno diplomatico e logistico ai nostri concittadini. Non da ultimo, non ho capito il motivo per cui rifiutate di accettare il fatto che abbiamo messo a disposizione fondi e medicinali per i nostri concittadini.

Il più recente, senatore Casini, è del 2010, quindi di qualche anno fa, mentre il più datato è addirittura del 1861. Quindi io le dico che, invece di gridare all'urgenza, farci tutti un esame di coscienza. Fatevi un esame di coscienza su quello che non avete fatto nelle scorse legislature per questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È facile mettersi delle spillette colorate oggi; ma nella scorsa legislatura abbiamo fatto poco e niente per quel Paese. Senatore Casini, faccia il bravo. Senatore Lucidi, torniamo ad oggi. LUCIDI *(M5S)*. Sì, torniamo ad oggi. Noi non stiamo sostenendo lo *status quo* in Venezuela; noi stiamo semplicemente dicendo quello che diciamo da sempre, cioè che rifiutiamo ogni tipo di ingerenza esterna, in virtù di quel principio di autodeterminazione che sempre abbiamo sostenuto. Democrazia è saper parlare e saper ascoltare. Ci sono stati sei interventi consecutivi, con un'educazione che mi è sembrata strana in quest'Aula. Concludiamo in bellezza.

non mi sorprende il fatto che, anche quando abbiamo citato la nostra vicinanza di comuni intenti con la Grecia, siano tutti "esplosi". Guarda un po'; pensiamo un po' a chi l'ha inventata, la democrazia. Dovrebbero riflettere anche su questo, questi signori. dal Gruppo PD).* Chiudo semplicemente ringraziando il Ministro e userò le parole del mio collega, senatore Ferrara, il quale mi suggerisce una cosa molto di buon senso (quello che secondo me a voi manca). La posizione dell'Italia è molto delicata: centinaia di migliaia di nostri connazionali rischiano di trovarsi coinvolti in un conflitto dagli esiti incerti. Questo ci impone ancora di più la massima responsabilità e moderazione, e non certo toni da ultrà, come abbiamo sentito in quest'Aula oggi e pochi giorni fa. Oggi noi non sappiamo cosa accadrà nel prossimo futuro in quel Paese, ma abbiamo in testa nomi e luoghi. Tutti li abbiamo in testa, questi nomi e luoghi, e sono: Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e Ucraina, solo per citarne alcuni. In nessuno di questi casi precedenti la ricetta degli Stati che vengono posti a guardia dei principi di democrazia e prosperità ha ottenuto gli effetti desiderati. Ovunque, purtroppo, le ingerenze esterne hanno scatenato sanguinose guerre civili che durano da anni, devastazioni delle infrastrutture e delle città, distruzione delle istituzioni e dell'ordine che, seppur precario, permetteva una vita sicuramente migliore rispetto a quella che è venuta dopo.

anche al Nord ci sono problemi, o ci potrebbero essere, per scelte scellerate. In questo caso mi riferisco al Piemonte, che solo di recente è uscito da un commissariamento della sanità. Nonostante i problemi che ci sono (nei giorni scorsi molte notizie parlavano di Pronto soccorso sovraffollati e pazienti costretti in barella per giorni), abbiamo però delle eccellenze riconosciute a livello non solo nazionale, ma europeo. Mi riferisco al polo materno-infantile del Sant'Anna e dell'ospedale Regina Margherita, attualmente confluiti nell'azienda unica della Città della salute con le Molinette, ed altri presidi della città di Torino. Ebbene, l'attuale governo regionale ha previsto di ricollocare tutte le strutture presso il futuro Parco della salute, che intende realizzare nell'area del Lingotto. Potrebbe anche essere una buona idea costruire una nuova struttura con degli edifici moderni e sicuri dove allocare il meglio della sanità torinese, se non fosse che negli anni questo progetto ha visto scendere il numero dei posti letto complessivi ed in particolare quelli dell'area materno-infantile, che passerebbero dagli attuali 656 a 284, con una riduzione superiore al 55 È inaccettabile pensare che tra qualche anno i cittadini torinesi debbano trovarsi nella condizione di non poter far nascere i propri figli nella loro città o che, una volta nati, debbano portarli altrove per ricevere cure indispensabili. Dopo aver assistito, negli ultimi anni, alla chiusura di ospedali e punti nascita, ora il Partito Democratico piemontese si appresta ad infliggere un ennesimo colpo alla sanità pubblica regionale, ma noi non ci stiamo. Il MoVimento 5 Stelle si è sempre si è sempre opposto a questa politica distruttiva e continuerà a farlo. Per questo segnalo a tutti i torinesi, e non solo a loro, che sono in corso iniziative per manifestare chiaramente al governatore Chiamparino e a tutto il PD la contrarietà a questo progetto devastante ed in particolare l'invito, questo sabato alle 15, in Piazza Castello alla manifestazione «Un fiocco per il Regina Margherita e il Sant'Anna» perché le eccellenze vanno difese, potenziate e non smantellate.

prendo periodicamente la parola per denunciare ed evidenziare, purtroppo, fatti criminosi di matrice mafiosa che avvengono a Foggia e nella sua provincia, dove opera da decenni quella che ormai è nota ovunque come la quarta mafia italiana. È una mafia feroce che ha un controllo pervicace del territorio e che incute un profondo timore tra i cittadini e gli operatori economici. Questo clima di vero e proprio terrore è finalizzato a perpetrare traffici di stupefacenti e di armi, nonché ad assoggettare gli operatori economici alle estorsioni, oltre ad altri delitti. Negli ultimi mesi, le indagini della magistratura e delle Forze dell'ordine hanno portato all'arresto di numerosi e apicali esponenti dei clan della città capoluogo, oltre ad altri arresti che hanno colpito i clan di San Severo e di Manfredonia. Ma ciononostante, o forse anche in conseguenza di questi arresti e quindi del conseguente vuoto di potere criminale, si sono verificati in queste ultime settimane ben sette attentati dinamitardi ai danni di attività commerciali, di cui ben tre negli ultimi sei giorni e l'ultimo la notte passata. La volontà criminale è chiara: prostrare psicologicamente la cittadinanza, incutere il terrore tra i commercianti al fine di poterli taglieggiare comodamente. Questi episodi fanno seguito a una lunga serie di bombe che volevano intimidire anche i Carabinieri, perché vi ricordo che ci sono stati nei mesi scorsi degli attentati a due carabinieri, uno a Cerignola e uno a Corato, o anche a dirigenti comunali: vi ricordo quello ai danni di un dirigente di Monte Sant'Angelo che è un Comune che era stato sciolto per mafia ed era tornato al voto. In questo momento stanno operando le commissioni di accesso a Manfredonia e a Cerignola per verificare eventuali infiltrazioni mafiose in queste amministrazioni. La situazione, come ho cercato di spiegarvi, è gravissima e credo sia arrivato il momento per lo Stato di mettere in campo tutti i presidi e anche gli uomini necessari a contrastare questa mafia feroce. È necessario, a nostro giudizio, istituire al più presto una sezione di corte d'appello a Foggia e della DDA e a questo scopo il MoVimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge di cui sono primo firmatario. È altresì necessario istituire una sezione dislocata della DIA, la direzione investigativa antimafia, come il MoVimento 5 Stelle chiede sin dal gennaio del 2016. Concludo facendo appello al Ministro dell'interno, al Governo e a tutte le forze politiche presenti nel Parlamento: chiedo a tutti voi di prendere atto di questa situazione gravissima e di concorrere all'adozione di tutti i provvedimenti del caso. Ogni giorno che passa è un giorno perso nel contrasto alle mafie, a queste feroci mafie foggiane, e ogni giorno che passa senza agire è un favore ai criminali. *(Applausi

Sono rammaricata per gli agricoltori, che rappresentano una categoria di lavoratori silenziosa, elemento portante dell'economia pugliese. Ferme restando le presunte responsabilità addebitabili alla Regione Puglia, occorre comunque trovare soluzioni alternative al fine di ristorarli dai danni subiti in tempi brevi, essendo stati danneggiati circa 90.000 ettari di aree agricole ubicate nelle province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia. Il settore oleario, nell'anno 2018, ha perso circa 117 117 milioni di euro di produzione lorda vendibile, con il conseguente degrado delle infrastrutture connesse a tale attività. Riconoscendo pertanto la sensibilità del Presidente del Senato, del ministro Centinaio e del presidente del Consiglio Conte, chiedo un autorevole intervento, al fine di superare definitivamente questa gravosa questione, a sostegno degli agricoltori. *(Applausi dal

Il Ministro si era impegnato a fare alcune cose, ma non sta succedendo niente e siamo arrivati al punto che i cittadini di quel quartiere hanno fatto un esposto per chiedere il sequestro di un intero condominio occupato